la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 27 settembre 2007. Oggi pomeriggio, sul decreto-legge in materia di sicurezza stradale e sull'omologo disegno di legge trasmesso dalla Camera avrà luogo la discussione generale congiunta, a conclusione della quale si passerà, nell'ordine, alla distinta trattazione dei due provvedimenti, tutto nell'ambito di un'unica ripartizione dei tempi, per complessive otto ore e trenta minuti. Nella giornata di domani, a conclusione dei provvedimenti in materia di sicurezza stradale, proseguirà l'esame del disegno di legge recante delega sugli enti di ricerca e della legge comunitaria. Sarà inoltre iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge in tema di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 settembre, avranno luogo comunicazioni del Governo sulla revoca e sostituzione di un componente del Consiglio d'amministrazione della RAI. Le proposte di risoluzione e le eventuali riformulazioni potranno essere presentate entro le ore 11 dello stesso giorno. I Gruppi avranno a disposizione dieci minuti ciascuno (quindici minuti al Gruppo misto) per la discussione generale e ulteriori dieci minuti per le dichiarazioni di voto (ugualmente quindici minuti al Gruppo misto). La trattazione della materia si concluderà pertanto entro la mattina di giovedì 20 settembre, anche oltre il consueto orario. Per la prossima settimana, a partire dalle ore 11 di martedì 25 settembre, il calendario prevede - oltre al seguito degli argomenti non conclusi - il rendiconto e l'assestamento del bilancio, la seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Senato, sul disegno di legge di modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte, nonché i disegni di legge relativi al reato di tortura, alle professioni sanitarie, allo sportello unico per le imprese e infine le ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione. Nella seduta pomeridiana di giovedì 27 settembre, sono previste interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*). A tal fine, i Gruppi sono invitati a segnalare per tempo alla Presidenza i possibili argomenti, ai fini della individuazione da parte della prossima Conferenza dei Capogruppo, da convocare martedì 25 settembre.

richiamare la sua attenzione e la sua sensibilità sulla circostanza che uno dei membri di questo Senato, che per giunta ne è il Vice presidente e quindi agli occhi dei cittadini rappresenta questa istituzione, ha proclamato "la marcia dei maiali" per stanare i credenti di altre religioni, in particolare gli islamici, che volessero avere un luogo di culto nella Repubblica italiana. Mi sembra, Presidente, che si tratti di un fatto grave, innanzi tutto perché l'opinione pubblica può essere indotta a credere che quel Vice presidente del Senato ci rappresenta, e vorrei che i colleghi che non si sentono rappresentati, ma che anzi sono imbarazzati e si vergognano

dichiarato da Umberto Bossi, che chiede di non comprare più prodotti italiani: un fatto non tanto di grave serietà quanto di inaudita novità, perché non esiste Paese al mondo che proclami il boicottaggio di se stesso. poi richiamare le dichiarazioni dell'ex sindaco Gentilini, il quale ha invitato - cito il «Corriere della Sera» di ieri - allo stupro della madre di un membro del Parlamento e del Governo; non sto esagerando, è scritto qui, signor Presidente, perché è troppo volgare per essere detta in quest'Aula, ma è stata pronunciata dal rappresentante politico di una parte che siede in quest'Aula.

senatore Colombo, noi dobbiamo sempre (per il Presidente è sempre un punto di grande attenzione) distinguere le cose politiche, anche forzate, da

un atteggiamento, rispetto alle cose più delicate, corrispondente alle responsabilità che il popolo italiano ci ha dato e quindi cercherò di essere molto attento su queste questioni.

Io le ho chiesto più volte, per conto mio e di 30 senatori, la pubblicazione di una decisione del Consiglio di Presidenza del Senato che riguarda la modifica della previdenza dei senatori.

Ora, i miei colleghi e io scopriamo dal giornale che l'indennità dei senatori è aumentata di circa 200 euro, noi non conosciamo assolutamente ancora il testo che regolamenta la previdenza e l'adeguamento dell'indennità perché ancora non è stato distribuito, nel contempo invece non riusciamo a difendere, con i cittadini e con gli elettori, la correttezza del nostro comportamento, perché non sappiamo che cosa c'è dentro questa documentazione. Signor Presidente, con il dovuto rispetto che le devo, dichiaro che da oggi adotterò, nelle forme e nei modi che riterrò più opportuni per correttezza nei confronti della mia Capogruppo e nei confronti suoi, la rinuncia formale a questo aumento. Prego i colleghi di prestare un attimo di attenzione, perché la risposta al punto toccato dal senatore Lusi è una cosa seria.

La finanziaria dell'anno scorso ha stabilito il taglio del 30 per cento degli aumenti in questi settori. Il Senato, dopo aver approvato il bilancio interno per il 2007, ha provveduto ad applicare la legge, che prevede un diritto individuale di tutti i senatori. Questo è il quadro, rispettando la legge; quindi, dobbiamo partire da questo. Si può prendere una decisione che in qualche modo modifichi questa situazione? C'è un modo solo, al di là delle rinunce individuali, che poi trovano la via che debbono trovare:

altrimenti, è capitato che momentanee sospensioni dell'erogazione dell'aumento siano state recuperate dopo, anche con gli arretrati. Dichiaro che il Consiglio di Presidenza, e comunque il Presidente, è disposto - come abbiamo già fatto per quanto riguarda la previdenza, compiendo un lavoro serio - a ragionare anche di questo. Raccomando questo ai senatori: in una materia così delicata, cui si intrecciano incertezze, non conoscenze e momenti non ordinati, il Senato - come sto dicendo - naturalmente con la Camera, vuole ritoccare questo punto (e sono disponibile a discuterne), deve porsi l'obiettivo di cambiare la legge che ci lega automaticamente a quell'andamento. È privo di senso il rifiutare, il decidere da solo. Io apro il confronto

credo che bisogna smetterla di fare demagogia su un tema così importante. Condivido completamente il suo ragionamento e vorrei dire al collega Lusi che, invece di chiedere oppure

i parlamentari. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP).* Noi dell'opposizione abbiamo votato contro l'aumento per i magistrati e, di conseguenza, contro l'aumento per i parlamentari; la maggioranza ha voluto votare a favore dell'aumento, se adesso ha complessi di colpa, se li risolva. Noi eravamo d'accordo prima; lo siamo adesso, ma il moralismo non lo accettiamo, specie se, quando vi è l'occasione, la si perde perché si deve ubbidire ad una corporazione esterna alla quale non si ha il coraggio di dire di no. *(Applausi e ora con questo dibattito perché la strada che ho indicato è l'unica possibile, poi vi possono essere scelte individuali. Quindi, è inutile continuare. Ribadisco la disponibilità del Senato a parlarne, ma la strada è quella, altrimenti non ne usciamo.

che è stata identificata come l'anti‑Welby. Lei ricorderà, signor Presidente, che anche in quest'Aula abbiamo discusso del caso di una persona per la quale si sono mobilitate persino autorità istituzionali per costringere qualcun altro a decretarne la morte, contro ogni logica derivante dal diritto naturale. Ma non è questa la questione. Presidente, io, come parlamentare, tento di essere giudizioso e presento interrogazioni su tali materie; pertanto, avrei potuto tranquillamente a fine seduta rivolgerle un sollecito. Quando, però, le interrogazioni cominciano ad accumularsi, vuol dire che su questi casi

quanto accaduto nei giorni scorsi rispetto alla polemica seguita alle parole del Papa in tema di eutanasia, vorrei raccomandare alla sua attenzione la necessità che il Ministro della salute si renda conto di quanto sta accadendo a Piacenza riguardo alle condizioni di salute di un cittadino italiano, Gian Piero Steccato, colto da ictus e afflitto della cosiddetta sindrome del chiavistello (sono andato a trovarlo personalmente e muove solo un polpastrello). Ebbene, si ha la sensazione che lo si voglia indurre a rassegnarsi ha la sensazione che lo si voglia indurre a rassegnarsi alla morte. È inaccettabile che in un Paese in cui un posto letto in ospedale costa allo Stato 516 euro al giorno una persona in quelle condizioni venga trattata con la miseria di 23 euro al giorno. Presidente, le chiedo di poter fare di tutto affinché il Ministro della salute prenda in considerazione tale questione: è inaccettabile che lo Stato spinga al desidero di morire delle persone. Siamo in presenza di una persona che chiede di essere aiutata a vivere e Gian Piero Steccato ha diritto di vivere.

dovrebbero prevenire o comunque portare a contenere questo fenomeno che, come lei, Presidente, sa benissimo, ha colpito anche il nostro Abruzzo, come tante altre Regioni italiane con vittime e danni enormi, e con rischi rilevanti per la vita dei cittadini. Su questo tema, passata l'estate, o meglio il momento più caldo dell'estate stessa, non ho ascoltato una

per prevenire fenomeni del genere o per reprimere i reati che di questi fenomeni sono spesso il frutto. Presidente, la mia è una richiesta che faccio in maniera accorata e credo che risponda al desiderio di tanti di noi perché abbiamo vissuto l'estate più drammatica della storia italiana, almeno per quanto riguarda la mia memoria storica.

di sensibilizzazione verso il Presidente del Consiglio, dal momento che tutto ciò che è stato votato in finanziaria a favore della Sicilia, ad oggi, non è stato attuato nonostante i proclami. Non parlo di promesse verbali, ma di tutto ciò che è stato votato in finanziaria.

Signor Presidente, volevo pregarla di chiedere al ministro Mussi di venire a riferire in Aula per un fatto molto grave che sta inquietando, sta allarmando tutti i ricercatori, i professori, i docenti

a svolgere la loro attività istituzionale. È un fatto gravissimo. È inutile parlare di rilancio del sistema della ricerca, di investimenti nel sistema universitario quando non si mettono a disposizione le risorse

Lo ha fatto consapevole della gravità della situazione che permane sulle nostre strade e della necessità di adeguare il codice della strada alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per tutti gli utenti della strada. A luglio abbiamo avviato rapidamente la discussione sul disegno di legge recante, appunto, disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, Atto Senato n. complesso provvedimento di 35 articoli, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Voglio ricordare che la Camera ha elaborato ed approvato un testo partendo da un disegno di legge del Governo presentato al Parlamento che è stato sostanzialmente confermato nei suoi contenuti, ma anche notevolmente ampliato con nuovi e numerosi articoli aggiuntivi. un testo ampio, sostanzialmente e di fatto confermato anche dalla nostra Commissione lavori pubblici, che però ha apportato diversi, importanti e positivi modifiche e miglioramenti a quel provvedimento. Nell'imminenza dell'esodo estivo, però, è sorta da parte del Governo la necessità di far entrare subito in vigore alcune parti del testo,

tra maggioranza, opposizione e Governo di procedere alla discussione e votazione prioritaria dei sei articoli, che sono poi diventati il testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto, ministri il 3 agosto, riferiti ai seguenti temi: disposizioni in materia di guida senza patente; limitazioni alla guida in particolare per i neopatentati; disposizioni in materia di velocità dei veicoli con sanzioni molto più robuste; disposizioni restrittive sull'uso dei cellulari durante la guida; maggiori sanzioni e restrizioni per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; infine - l'ultimo articolo - norme atte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di ebbrezza. Voglio ribadire che il confronto in Commissione su questi articoli è stato molto accurato e costruttivo ed è stato grazie all'impegno naturalmente della maggioranza ma anche e soprattutto dell'opposizione, che ha assicurato un dialogo continuo, insieme al Governo, se siamo arrivati congiuntamente a questo importante risultato. La Commissione - maggioranza e opposizione concordi - ha sempre ritenuto, d'intesa con il Governo, che fosse necessario puntare ad una rapida approvazione del disegno di legge, lo ricordo - include anche i sei articoli inseriti nel decreto-legge n. 117 al nostro esame, perché di portata più ampia e perché affronta i diversi aspetti di prevenzione, tecnologie, norme e repressione che il tema della sicurezza stradale richiede. Per questa ragione, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la Commissione ha proseguito il proprio lavoro completando l'esame del disegno di legge e dei numerosi emendamenti presentati, arrivando la scorsa settimana alla sua approvazione. Per le medesime Per le medesime ragioni, perché abbiamo ritenuto che quello fosse il provvedimento prioritario già in corso come concordato, non siamo stati nelle condizioni di concludere l'approvazione del decreto-legge,

proprio per evitare rischi anche solo potenziali di vuoti normativi in materia di grande delicatezza sociale, giuridica e penale, e di proseguire, dopo dopo il voto su tale provvedimento, alla disamina dell'articolato del disegno di legge affinché i due testi siano coordinati ed unitari e siano inviati in modo immediato all'altro ramo del Parlamento. Sono certa che gli esponenti dell'opposizione, che hanno assicurato in Commissione un contributo concreto ed assai responsabile per l'approvazione del provvedimento, sanno e sapranno comprendere le ragioni della necessità di approvare in quest'Aula entrambi i provvedimenti. Naturalmente siamo tutti consapevoli che, nonostante i miglioramenti apportati dal lavoro in Commissione, tenendo conto di altre modifiche che saranno poste all'attenzione dell'Aula, sostanzialmente in buona parte già concordate, dovremo continuare ad intervenire - lo dico in particolare al Governo - su due questioni che il provvedimento non assolve nella sua interezza: l'attuazione del piano sulla sicurezza stradale e l'aumento dei numeri dei controlli sulla strada. Infatti, solo da questo deriverà poi una piena ed efficace attuazione delle nuove norme che stiamo predisponendo;

Quindi, nel riferire sull'andamento dei lavori della Commissione, ho rappresentato la complessità di un *iter* che ha assicurato un'articolata disamina del provvedimento - e quindi il pieno rispetto delle prerogative della Commissione lavori pubblici

Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento in approvazione costituisce una prima importante risposta ad un bisogno di sicurezza particolarmente avvertito nel nostro Paese. Gli oltre 5.500 morti che annualmente continuano a registrarsi, insieme agli oltre 25.000 feriti con conseguenze permanenti, derivanti dagli oltre 300.000 incidenti, ci parlano con tutta evidenza di una realtà che non è assolutamente fuori luogo paragonare a uno stato di guerra. E a poco vale il fatto che negli ultimi anni questo Paese ha intrapreso un'apprezzabile riduzione delle morti per incidenti stradali, dato che rimaniamo ancora ben distanti dall'obiettivo comunitario che abbiamo assunto, quello di dimezzare il numero di morti e incidenti stradali registrati nel 2000 entro il 2010. risultati comunque sono il frutto non casuale di provvedimenti che in questi anni hanno dispiegato la loro efficacia: penso soprattutto al provvedimento istitutivo della patente a punti, ma più in generale anche a quei provvedimenti che hanno disciplinato l'uso del cellulare, l'obbligatorietà del casco o l'uso delle cinture che hanno consentito di salvare migliaia di vite umane. La sicurezza stradale costituisce da tempo, infatti, un tema particolarmente caldo nel nostro Paese e un ambito legislativo privilegiato di intervento, sia per adeguare il nostro ordinamento alle direttive comunitarie, sia per concorrere all'obiettivo europeo sopra richiamato; un obiettivo senz'altro ambizioso, su cui il nostro Paese mostra di marcare il passo, ma proprio per l'importanza che riveste non consente assolutamente incertezze o ripensamenti. È piuttosto un altro concetto di sicurezza, un'altra cultura della sicurezza stradale

un'altra cultura della sicurezza stradale quella che occorre affermare per fare il salto di qualità necessario. Gli esempi in Europa, da questo punto di vista - come sappiamo - non mancano e ad essi è spesso utile riferirsi. Ce ne siamo resi conto una volta di più nel lavoro che ha impegnato la Commissione. Mi sia consentito per questo di rivolgere un particolare apprezzamento e ringraziamento ai colleghi dell'opposizione che hanno reso possibile, oltre ad un proficuo confronto, sempre utile, anche la ricerca di risposte e di soluzioni condivise a problemi e questioni di particolare delicatezza che investono la sicurezza, ma anche le abitudini di vita di milioni di nostri concittadini. Un ringraziamento doveroso anche al Ministro che ha seguito insieme agli uffici e ai suoi più stretti collaboratori tutto l'*iter* dei lavori dell'8a Commissione, manifestando una disponibilità ed un'apertura non ordinarie e che si sono rilevate quanto di più necessario occorre, su temi tanto delicati e importanti come quello della sicurezza stradale, dove in gioco vi sono - lo ripeto - migliaia di vite umane ogni anno. Sono altresì convinto che ulteriori miglioramenti potranno essere apportati anche durante la discussione che ci accingiamo ad intraprendere in Aula e sono comunque certo che dal nostro dibattito potrà venire un contributo importante per la futura delega al Governo di revisione del codice della strada, prevista nel provvedimento in esame. Il tema centrale, a mio avviso, è quello costituito dalla necessità di intraprendere la strada per affermare una nuova cultura della sicurezza, fondata su tre pilastri essenziali: una una prevenzione e un'educazione stradale particolarmente rivolta ai giovani e segnatamente presente nelle scuole di ogni ordine grado in ragione specie dei comportamenti alla guida sui quali è particolarmente urgente intervenire con un'inversione di rotta consapevole da parte degli utenti della strada; un quadro normativo e sanzionatorio adeguato, sia all'evoluzione che la tecnologia ha registrato in questi anni, sia a dare certezza alla pena prevista per ogni violazione. Infine, ma non ultimo per importanza, una maggiore intensificazione dei controlli e degli accertamenti che collocano ancora il nostro Paese molto indietro rispetto agli *standard* europei. Una cultura della sicurezza stradale che deve affermarsi a partire, in primo luogo, anche dalle discussioni in famiglia e nella scuola, le prime agenzie formative nella vita di un giovane, le uniche in grado di stimolare una coscienza critica dell'individuo, tanto necessaria quando il gruppo dei coetanei successivamente, nel processo di crescita e di affermazione della propria autonomia, tenderà a prevalere nell'orientamento dei comportamenti, mettendo a dura prova quei precetti basilari - verrebbe da dire di buon senso - assunti fino a quel momento come valori di riferimento. Una cultura della sicurezza stradale che deve affermarsi, quindi, non con proclami o con eventi sensazionali, ma piuttosto con esempi quotidiani del rispetto, anche da parte dell'adulto, sia esso genitore o insegnante, delle norme più elementari del codice della strada. Anche in questo caso potremmo dire che ciò che occorre è il ripristino di un senso del rispetto della legalità di cui spesso noi avvertiamo la fragilità. Nelle settimane che ci stanno alle spalle è impresso in tutti noi il ricordo di una scia di sangue consumata sulle strade del nostro Paese, di particolare drammaticità e gravità. Giustamente, i mezzi di informazione hanno amplificato l'attenzione sulle cause, sulle dinamiche e sulle conseguenze che hanno provocato queste tragedie. Amplificati, giustamente, sono stati i comportamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione a causa di sostanze stupefacenti che, nell'ambito della causa principale degli incidenti costituita dall'eccesso di velocità, ha rivestito negli ultimi anni sempre più importanza e significato. Di fronte ai nostri occhi vi è uno scenario che probabilmente non si risolve soltanto con le pur necessarie restrizioni normative e gli inasprimenti sanzionatori, ma che richiede un intervento più in profondità nella nostra società, a partire dai luoghi di aggregazione e di incontro delle giovani generazioni, e richiede obiettivi più alti per suscitare condivisione nelle coscienze di ognuno. Talvolta, invece, il nostro complesso sistema di regole, le nostre migliori intenzioni e i nostri condivisibilissimi obiettivi sembrano infrangersi e risultano come impotenti di fronte a quelle che ormai da anni definiamo "le stragi del sabato sera" e che ogni anno moltiplicano i propri effetti quasi come se rispondessero ad un altro sistema di valori. Il punto è che in questi anni la tecnologia ha fatto indubbiamente passi da gigante, migliorando le prestazioni e gli *standard* di sicurezza dei veicoli, migliorando la sicurezza e le infrastrutture stradali, ma non altrettanti passi corrispondenti sono stati fatti sullo stile dei comportamenti di guida. Banalizzando potremmo dire che le coscienze degli individui sono risultate meno flessibili e meno malleabili della tecnologia che abbiamo sviluppato. In questo senso, probabilmente, la nuova frontiera dell'applicazione tecnologica, per la sicurezza stradale come per altri ambiti, non può non essere la sua applicazione al controllo dello stato psicofisico e alle condizioni della persona alla guida: la macchina che controllo l'uomo e lo abilita alla guida! Sta forse in questo paradosso il segno dei tempi in cui le stridenti contraddizioni che si manifestano si potranno risolvere in un futuro solo ribaltando il paradigma fino ad oggi noto. Il provvedimento oggi in esame in quest'Aula ha conosciuto nei lavori della Commissione sostanzialmente due fasi: la prima, che ha coinciso con la chiusura dell'attività parlamentare in occasione del riposo estivo, ha consentito al Governo, con lo stralcio, ricordato dalla Presidente, dei sei articoli che rivestivano nell'articolato carattere di particolare urgenza, di emanare il decreto-legge per fronteggiare quella che già si annunciava un'estate all'insegna dell'emergenza sicurezza. I sei articoli hanno riguardato: la guida senza patente, alcune limitazioni alla guida per i neopatentati, una nuova articolazione degli eccessi di velocità, una nuova disciplina nell'uso del cellulare e una revisione normativa della guida in stato di ebbrezza alcolica o in condizione di alterazione a causa di sostanze stupefacenti. È sicuramente presto per dare un giudizio compiuto sugli effetti che questi provvedimenti hanno prodotto, e sicuramente i dati a disposizione non consentono un presupposto di attendibilità. Certo è che comunque è riscontrabile una maggiore attività nei controlli sulle strade e negli accertamenti realizzati emergono tratti particolarmente inquietanti negli stili e nei comportamenti di guida in specie riferiti ai giovani, dati che comunque ci incoraggiano nel proseguire un'azione che non può conoscere cedimenti o incertezze. La seconda fase è quella attuale che vede, alla riapertura dei lavori parlamentari, il provvedimento in Aula già interamente esaminato della Commissione, tenendo fede ad un impegno assunto prima della pausa estiva. La buona politica, attesa e voluta dai cittadini, mi permetto di dire in maniera sommessa e con la massima umiltà, è anche questa: quella politica, cioè, che di fronte a problemi concreti, drammatici e quotidiani come quelli della sicurezza stradale, che distruggono la vita di migliaia di famiglie, riconosce e sa anteporre l'interesse generale della collettività rispetto al legittimo interesse del proprio tornaconto politico. Quella politica che in queste situazioni sa stringere patti per quei superiori interessi e li mantiene, indipendentemente dalle contingenze politiche del momento. In questo senso, mi preme dare atto di un comportamento ineccepibile in Commissione da parte dei colleghi dell'opposizione, che spero si possa mantenere anche in Aula. Il provvedimento esaminato in Commissione e proposto per l'Aula ci consente, tra l'altro, di apportare significativi miglioramenti anche ad alcune lacune manifestate nell'applicazione del decreto-legge, come per esempio la depenalizzazione del rifiuto circa l'accertamento delle proprie condizioni psicofisiche, dando luogo ad una procedura elusiva del tutto intollerabile, o come l'eccessiva restrizione delle limitazioni di guida per i neopatentati, che ha suscitato preoccupazioni e contrarietà in molte famiglie italiane, che pure ne comprendevano le ragioni. Il testo giunto in Aula e sottoposto alla discussione si compone così di 38 articoli, che vanno a costituire un articolato normativo organico in grado di apportare significative correzioni al codice della strada, in ragione delle stringenti necessità, ma anche di definire ambiti precisi di delega al Governo, per una sua necessaria rivisitazione complessiva, tesa in buona sostanza ad armonizzarlo con le direttive comunitarie intervenute, a semplificarlo opportunamente e a disciplinarne nuovi ambiti di applicazione. È opportuno inoltre segnalare che il provvedimento in esame ha la necessità di concludere il suo *iter* di approvazione, come è stato ricordato, entro il 3 ottobre, termine di decadenza del decreto emanato dal Governo, consentendo per quella data la necessaria approvazione in terza lettura ai colleghi della Camera dei deputati, onde evitare uno sconveniente vuoto legislativo in coincidenza della decadenza del decreto stesso. In questo senso, è da ravvisare che, nonostante le correzioni e gli apporti intervenuti in Commissione, il testo licenziato dalla Camera ed approvato a larga maggioranza, mantiene integralmente la sua struttura e la sua identità originaria. Possiamo quindi dire che nella sostanza è stato sì modificato, ma non stravolto. Gli articoli centrali del provvedimento rimangono costituiti dall'articolo 12, che disciplina le sanzioni previste per gli eccessi di velocità; dall'articolo 16, che configura - con altri ad esso affini - un nuovo quadro normativo della guida in condizioni di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; dall'articolo 31, oggetto di delega al Governo per riformare il codice della strada. Queste, comunque, sono le principali modifiche intervenute, che riassumo sinteticamente per brevità. All'articolo 1, sono state previste norme di inasprimento sanzionatorio in materia di regolamentazione della circolazione nei centri urbani, finalizzate alla riduzione degli inquinamenti atmosferici ed acustici. È stato abrogato l'ex articolo 2, che disciplinava la guida accompagnata e che prevedeva il rilascio del foglio rosa ai sedicenni a particolari condizioni, anche se non ne viene in futuro preclusa la previsione, diventando oggetto specifico di delega al Governo nella rivisitazione del codice della strada. È stato inoltre previsto, sempre nell'ambito dell'esercizio della delega, l'obbligo dei 16 anni per la guida dei quadricicli leggeri, oggi impropriamente assimilati ai ciclomotori. Ancora, nell'esercizio della delega, viene previsto il recepimento anticipato della direttiva comunitaria che va a disciplinare l'armonizzazione in materia di patenti di guida. All'articolo 5, sono introdotte nuove misure di limitazione della guida per i neopatentati. All'articolo 12, viene introdotto il divieto di trasporto su motocicli e ciclomotori a due ruote di minori di quattro anni. All'articolo 13, sono previste ulteriori limitazioni nell'esenzione dal divieto dell'uso del cellulare alla guida, restringendolo alle sole Forze armate e ai Corpi di polizia, prevedendo l'inasprimento sanzionatorio della sospensione della patente in caso di recidiva per gli altri

All'articolo 16, viene prevista un'ulteriore fascia dei tassi alcolemici riscontrabili alla guida, consentendo di graduare maggiormente le pene dallo stato di ebbrezza a quello di manifesta ubriachezza. All'articolo 24, sono previste misure sanzionatorie per quei locali che svolgono attività di spettacolo congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche e non ottemperano alle nuove disposizioni di informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. Di grande importanza è l'introduzione all'articolo 28 della previsione di destinare un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento al potenziamento dei servizi di controllo sulle strade, tema centrale per la realtà del nostro Paese. Più in generale, quindi, le norme del codice della strada modificate vanno a restringere il quadro normativo e a inasprire i termini sanzionatori riferiti agli eccessi di velocità e ai comportamenti di guida alterati dal punto di vista delle condizioni psicofisiche, fenomeni che - come sappiamo - costituiscono la prima causa di morte sulle strade italiane e purtroppo la prima causa di morte per i giovani sotto i 24 anni. Come riflessioni conclusive, anche in previsione di esercizio delle delega al Governo, vi sarebbe da aggiungere la questione di un maggiore raccordo con gli organi di governo delle istituzioni locali, anche in ragione di una differenziazione che si registra nell'attività di controllo sul territorio nazionale, ma anche per il fatto che che la maggior parte dell'incidenza dei morti sulla strada avviene proprio in ambito urbano. In ultimo, e concludo, vi è l'incremento esponenziale registrato dal nostro Paese negli ultimi decenni in termini di parco veicolare circolante, che ci vede ai primi posti della classifica mondiale e che costituisce causa non secondaria anche nell'aumento degli incidenti registrati, questioni che spingono con forza a promuovere e incentivare una maggiore diversificazione modale nelle politiche della mobilità riferita alle persone e alle merci.

sul quale troppo spesso c'è superficialità anche da parte degli operatori dell'informazione e nello scrivere le norme. Probabilmente, la concitazione nella necessità di rispondere alla pubblica opinione rischia di farci commettere degli errori. degli errori. Ministro, non ricordo se la questione che sarà oggetto di un emendamento specifico è frutto solo del lavoro del legislatore in Commissione o proviene direttamente dal Ministero; mi riferisco alla questione che ho segnalato alla pubblica opinione proprio nella giornata di ieri e che riproporrò in termini emendativi e soppressivi, riguardante una specie di indulto preventivo che si applicherebbe alla sicurezza stradale. La questione, Presidente, è la seguente. Giustamente si

Qui non ci si riferisce al danno che si provoca, perché per fortuna per il danno esiste altro tipo di sanzioni, ma alla semplice guida di un veicolo senza la patente; se si prevede l'arresto - come è scritto nella norma - non si capisce perché lo si debba prevedere la seconda volta e non la prima,

perché credo che non dobbiamo dare all'opinione pubblica l'immagine di un Parlamento che dice che la prima volta la si fa franca e alla seconda scatta l'arresto. Altre questioni sottoporremo all'attenzione dell'Aula, del relatore e del Ministro

Dette questioni saranno oggetto di cinque ulteriori emendamenti che cito qui per materia, riservandomi di intervenire poi nel corso della discussione.

perché noi dobbiamo evitare che i cittadini che con una automobile distruggono il patrimonio pubblico possano farla franca. Questo sarà oggetto di emendamenti riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Altra questione che intendiamo sollevare nell'ambito di questo provvedimento è la necessità di restituire al magistrato del tribunale una competenza che è stata devoluta al giudice onorario. Non sfuggirà al Ministro e ai relatori che si tratta di una Su tali vicende non si giudica solamente secondo cognizioni di carattere giuridico dato che effetti sociologici e psicologici concorrono a creare il giudizio del magistrato, giudizio che evidentemente non può essere affidato al giudice onorario, di per sé delegato dalla legislazione ai microconflitti e non a questioni di una rilevanza così specifica. Un'altra questione su cui vorrei soffermare l'attenzione, partendo da una valutazione positiva della norma in oggetto,

che può servire anche a risolvere le problematiche che ho visto segnalate anche in altri emendamenti e in alcuni ordini del giorno, ma che non ho visto approfondire in maniera specifica con una proposta normativa. *(Applausi

condivide pienamente l'obiettivo a cui mirano il Governo e il Parlamento con questo disegno di legge, vale a dire limitare gli incidenti stradali e dare più sicurezza ai cittadini sulle strade. evidenziare un particolare problema che si presenta soprattutto d'estate sulle strade di montagna che sono tormentate sempre di più

risposta alla nostra richiesta di controllare meglio sia i veicoli stessi, spesso truccati, che la velocità e il rumore nei paesi. Detto questo

infatti che se i controlli fossero effettuati in modo equo su tutto il territorio nazionale,

c'è una rete molto fitta e una severità incredibile nel controllo, nella sanzione e nella sua applicazione. Adesso, annunciando

che prevede multe molto aspre, devo porre una domanda: può darsi che per un parlamentare o per qualcuno che può permetterselo una multa di mille, duemila, tremila euro non faccia tanto male; farà male al portafoglio, ma non lo rovina;

che mille euro per uno che guadagna bene e mille euro per una famiglia, invece, bisognosa fanno una grande differenza: sono, da una parte, un dolore al portafoglio e, dall'altra, una strage completa.

perché costringere i nostri figli a guidare automobili che possono essere schiacciate come le scatolette delle sardine mi fa veramente paura.

che le misure più efficaci dovrebbero essere quelle preventive, le misure sociali e soprattutto le misure educative nelle scuole. A tal fine, abbiamo presentato l'ordine del giorno G103 che illustro molto brevemente. In esso praticamente si chiede che un articolo già vigente nel codice della strada, cioè il 230, trovi effettiva applicazione, al fine di svolgere un'attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado

di sfruttare meglio i mezzi a disposizione del Fondo nazionale per la sicurezza, che potrebbero essere messi a disposizione, come chiediamo con questo ordine del giorno, anche dei Comuni e degli enti locali che si attivano

l'uso delle carrozzelle per i portatori di *handicap*. Siamo stati avvertiti dalle associazioni di portatori di *handicap* che il codice della strada, così come si presenta, non tanto per la legge in sé ma per i regolamenti che ne sono

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha contribuito ampiamente,

signor Presidente, che questa sia una anomalia che questo Parlamento deve cominciare a denunciare. Sono da tanti anni in Parlamento e sinceramente non mi è mai capitato un fatto anomalo di questo genere. Dico anomalo perché, mentre noi stasera o domani mattina arriveremo alla conversione del decreto-legge così come presentato dal Governo, c'è l'intesa col Governo di apportare in Commissione una serie di modifiche sull'analogo disegno Mi sembra un fatto un po' schizofrenico: sarebbe stato molto più serio che il decreto fosse stato lasciato decadere e, con gli emendamenti che modificavano una parte del decreto medesimo, arrivare ad un disegno di legge organico più complessivo.

proprio per questa anomalia incomprensibile in questo Parlamento), vengo al merito del disegno di legge e anche del decreto-legge. Vede, signor Presidente, oggi potremmo definire il decreto e il disegno di legge un "multometro", un sistema di multe aggravate pesanti; non

bisogna dire che la polizia stradale deve avere più personale, più mezzi, bisogna mettere segnali, barriere, eccetera. Poco ci interessa, caro Ministro, che poi accolga il nostro ordine del giorno, sottoscritto anche dagli altri Gruppi, che il Governo si impegnerà a trovare i soldi: gli ordini del giorno sono come i sigari di Cavour, non si negano a nessuno. Ma non basta: prevenzione vuol dire - proposta respinta, che abbiamo ripresentato in quest'Aula e che spero i colleghi approvino l'obbligo dell'insegnamento nelle scuole dell'educazione stradale. Continuiamo a parlare di educazione stradale, altrimenti, come ho detto più volte in Commissione, cambiamo il titolo, chiamiamola legge delle quattro ruote, delle automobili. Se questo è il codice della strada, deve esserlo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Questo si fa cominciando dalle scuole elementari, insegnando ai ragazzi l'educazione civica.

quello delle pene accessorie cioè dei lavori socialmente utili. Ci si viene a dire che ciò è in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione

perché come sulla scuola non andiamo in contrasto con il Ministro della pubblica istruzione (per carità, non entriamo in casa d'altri, rendendo obbligatoria un'ora alla settimana di insegnamento del codice della strada), sul problema delle pene accessorie non andiamo a modificare il codice penale, perché entriamo in contrasto con il Guardasigilli, eccetera.

è agli arresti domiciliari, dopo pochi giorni; un pluriomicida, perché nel nostro codice si chiama omicidio colposo. Abbiamo proposto

Penso alle famiglie dei morti, signor Ministro. Allora noi dobbiamo prevenire, insegnare ai nostri ragazzi cos'è il codice della strada, se vanno in bicicletta, a piedi o in motocicletta. Basti vedere come circolano i motociclisti e i ciclisti

Signor Presidente, Ministro, la triste cronaca degli incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade ha riportato il tema della sicurezza stradale al centro del nostro dibattito politico, imponendo l'adozione di iniziative concrete a tutela della vita dei cittadini, anche alla luce dell'impegno assunto dall'Italia nell'Unione Europea, quello di dimezzare entro il 2010 il numero degli incidenti. Gli ultimi dati statistici evidenziano come in Italia ogni anno si verifichino circa 225.000 incidenti stradali, 5.426 decessi, oltre 300.000 feriti, con il 30 per cento delle vittime di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Sono numeri questi, signor Ministro, che, oltre a tenerci lontano da quei Paesi europei che vantano i più alti livelli di sicurezza stradale (Regno Unito, Svezia e Olanda), mettono in evidenza l'urgenza di adottare azioni più forti ed incisive in grado di migliorare e rafforzare la normativa posta a tutela della sicurezza stradale. Certamente il disegno di legge del Governo che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula è il frutto di un intenso lavoro svolto in Commissione. Un lavoro che, avendo coinvolto tutti i Gruppi parlamentari, offre anche importanti spunti su cui impostare rilevanti azioni finalizzate alla drastica riduzione degli incidenti stradali. Ci preme tuttavia denunciare che l'opportunità di realizzare concrete iniziative nel campo della sicurezza stradale ha trovato in questi mesi il suo limite più grande nell'evidente mancanza di volontà di questa maggioranza di voler rendere seriamente operative ed efficaci le misure contenute nel disegno di legge in esame, negando quelle risorse finanziarie che sarebbero state necessarie a dare consistenza alle azioni prospettate. Pertanto, se da una parte possiamo ritenerci soddisfatti dell'approvazione di alcuni importanti emendamenti presentati dal nostro Gruppo, riferendomi anche alle misure volte alla salvaguardia della vita dei giovani che sempre più spesso rimangono coinvolti in gravissimi incidenti stradali, dall'altra lamentiamo il fatto che queste misure non siano state adeguatamente supportate da opportune risorse in grado di renderle immediatamente efficaci. Ad esempio, la previsione dell'incremento del numero di controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine, che peraltro deriva dall'approvazione di un emendamento del nostro movimento della Lega Nord, pur rappresentando un'iniziativa efficace per contrastare l'elevato numero di morti nelle nostre strade, rischia di rimanere non applicata per le scarse risorse finanziarie disponibili. Proprio per quanto concerne i controlli nei confronti di chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, è opportuno ricordare che l'uso di tali sostanze è tra le principali cause dei sinistri. Tuttavia, nel periodo 2002-2004 solo il 3 per cento dei patentati italiani è stato controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi. In Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli l'anno, in Spagna circa 3-4 milioni, mentre in Italia i controlli sono appena 200.000. Oltretutto, bisogna considerare che l'uso smodato di sostanze alcoliche e di stupefacenti non rappresenta più un fatto occasionale, ma sta diventando una vera e propria piaga. Il nostro Gruppo ha quindi presentato alcuni emendamenti finalizzati all'inasprimento delle sanzioni accessorie nei casi di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, i quali sono stati accolti nel testo in esame. Tuttavia, riteniamo che tali misure debbano essere supportate da ulteriori interventi di natura penale che prevedano, da una parte, l'introduzione del reato di omicidio doloso per chi uccide guidando sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e dall'altra, l'applicazione di pene certe e più stringenti per chi commette i suddetti reati. In questa direzione vanno gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo in Aula, la cui approvazione permetterà di compiere importanti passi in avanti, indispensabili per contrastare l'elevato numero di incidenti mortali sulle nostre strade. Muovendo dalla necessità di affiancare ai suddetti interventi altre misure di natura maggiormente preventiva, il Gruppo ha poi presentato alcuni emendamenti che perseguono l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza stradale attraverso l'adozione di importanti iniziative quali l'obbligo per le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci di esporre al pubblico la lista dei medicinali che riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché il divieto di fumo durante la guida, anche per tutelare la salute dei cittadini ed in particolare le categorie più deboli, ed infine il finanziamento di corsi di educazione stradale nelle scuole. In particolare, auspichiamo l'approvazione di quest'ultimo emendamento, sostenuto fra l'altro anche da altri senatori dell'opposizione, di poter realizzare una seria prevenzione degli incidenti stradali permettendo ai giovani utenti della strada di maturare una cultura della sicurezza stradale, che sia poi in grado di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili durante la guida. Infine, a completamento dell'importante azione di rinnovamento portata avanti dal nostro Gruppo sulle norme poste a tutela della sicurezza stradale, è stata ravvisata la necessità di prevedere, tra i princìpi e i criteri direttivi della legge delega per la riforma del codice della strada, la revisione della normativa in materia di patenti di guida agli extracomunitari. Infatti, secondo le statistiche quasi una patente nuova su cinque è conseguita da immigrati. Anche se gli stranieri detengono il 5,34 per cento delle patenti italiane, essi sono responsabili del 6,08 per cento delle infrazioni, incidendo negativamente sui livelli di sicurezza stradale. Pertanto, ci auguriamo che anche in questo ambito possano giungere da parte della maggioranza e del Governo dei segnali positivi al fine di creare un sistema di regole maggiormente rigorose nei confronti di extracomunitari che intendono circolare in Italia con patenti rilasciate da Paesi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto comunque degli Accordi e delle convenzioni internazionali cui il nostro Paese aderisce. Concludendo, auspichiamo che gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo siano attentamente valutati durante l'esame del provvedimento in Aula, in quanto riteniamo che gli stessi possano fornire risposte maggiormente concrete, rispetto a quelle fin qui adottate, su un problema così importante come quello della sicurezza sulle strade e della tutela della vita umana: un po' di coraggio in più, mi permetta di dirlo, signor Ministro, da parte di tutti noi per non vanificare le aspettative dei nostri cittadini.

limitazioni alla guida in particolare per i neopatentati, le disposizioni in materia di velocità dei veicoli con le relative sanzioni, le disposizioni sull'uso dei cellulari durante la guida, le sanzioni e le restrizioni per la guida in stato di ebbrezza

di un dibattito proficuo e sereno. Il Ministro, la Presidente e il relatore sanno che però le nostre posizioni in merito erano e restano distinte e distanti, come abbiamo spiegato argomentando nel dettaglio la nostra posizione in sede di dibattito in Commissione e come intendiamo fare anche qui.

ai massicci spostamenti di auto sulle strade per le meritate vacanze. Non so, signor Ministro, quale sia il bilancio finale riguardante la sicurezza stradale nel mese d'agosto e in questo primo stralcio del mese di settembre, ma ho la sensazione che il decreto non abbia migliorato granché la situazione della sicurezza stradale, né abbia contribuito sensibilmente alla riduzione degli incidenti e dei decessi. Cercherò la sintesi, che ho già utilizzato peraltro in Commissione, per ribadire la posizione di Alleanza Nazionale. Siamo convinti che non si produca sicurezza solo elevando le sanzioni siamo convinti della necessità di operare su più fronti coniugandoli tra loro. Pensiamo a pene rapportate alla gravità dell'infrazione; alla modifica di comportamenti errati; ad una più fitta rete di controlli idonei a far rispettare le leggi e i divieti che già esistono. Tutto ciò ed altro concorre a creare la sicurezza stradale. In questo provvedimento abbiamo ravvisato una sorta di sindrome emotiva, che mai dovrebbe colpire il legislatore di qualsiasi colore. Allora, sulla questione ebbri o ubriachi, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'azione di droga è un problema serissimo, come lo è l'ignoranza della segnaletica o il mancato rispetto delle più elementari norme della convivenza sulle strade, ma l'inasprimento delle sanzioni non è tutto. Forse dobbiamo avere più coraggio. Noi lo avremmo avuto e avremmo potuto dire, prima di elevare le sanzioni che colpiscono chi si mette al volante alterato: o bevi o guidi. L'alternativa è certamente drastica, signor Ministro, ma potrebbe essere efficace, se opportunamente trattata sotto il profilo culturale, vorrei dire anche sotto il profilo pedagogico, e non solo per i giovani. Voi elevate le sanzioni, prevedete l'arresto per tutti,

Ripeto: sarebbe più opportuno dire «o bevi o guidi ». È un controsenso. Se consentite di bere, dovete consentire anche la gradualità delle sanzioni: quella del «o bevi, o guidi» è una scelta coraggiosa che non concederebbe nulla all'ambiguità delle percentuali di alcol o di altre sostanze nel sangue. Lo stesso vale per gli stupefacenti: sarebbe più coraggioso dire che non è mai lecito drogarsi, come Alleanza Nazionale sostiene da tempo e, comunque, a maggior ragione, prima di mettersi alla guida di qualsiasi mezzo. Ci domandiamo: ci sarà una differenza tra chi beve a cena un bicchiere di vino e chi si mette ubriaco alla guida? Questa differenza la prevede anche il codice della strada. Ci sarà questa differenza anche per quanto concerne le sanzioni? La risposta è negativa. Mi meraviglio sentire colleghi solitamente razionali che ritengono che aumentando le pene diminuiscano i reati e, quindi, in questo caso, gli incidenti. Si contrasta un reato se lo si persegue effettivamente, cioè attraverso un elevato numero di controlli che consentano alle forze di polizia di attribuire un significato anche educativo e preventivo al loro intervento. Non si può, a fronte di un risibile numero di controlli, di una scarsa politica di prevenzione e di educazione, affidarsi solo alla repressione, che - intendiamoci - è necessaria, ma non è ancora sufficiente. Sorrido quando leggo che bisogna imporre a tutti gli automobilisti un etilometro - come qualche collega ha proposto - da conservare in auto. Sorrido quando leggo statistiche per cui in Italia si può incorrere in un controllo di questo genere ogni 175 anni, signor Ministro. Sorrido amaramente se penso che nell'arco decennale della validità di una patente l'automobilista può ammalarsi, anche gravemente, e può dover assumere farmaci molto particolari, paradossalmente molto più pericolosi del classico bicchiere di vino. Pertanto, occorre un nuovo modello culturale. Occorre introdurre nuovi modelli culturali già nelle scuole per educare le giovani generazioni al valore della vita e al rispetto per gli altri e trasferire tali princìpi anche sulle strade. Occorre sensibilizzare tutti, ma soprattutto i giovanissimi, circa i rischi che derivano da un'eccessiva confidenza con gli alcolici o da un qualsiasi approccio con droghe. Forse, sarebbe opportuno ipotizzare - come già qualcuno ha ricordato - nell'educazione civica insegnata a scuola anche un piccolo capitolo dedicato all'educazione stradale.

Non intendiamo criminalizzare nessuno, ma vorremmo evitare l'ipocrisia, perché buona parte delle cosiddette stragi del sabato sera originano proprio da qui, cioè dalla distribuzione incontrollata di sostanze alcoliche ai giovani nei bar, nei pub e nelle discoteche. In questa materia abbiamo tanto da lavorare e mi riferisco soprattutto alla prassi, appunto, di vendere i superalcolici ai minorenni o a giovani che sono già evidentemente alterati. Prevedere per i gestori dei locali di intrattenimento l'esposizione di una tabella informativa sulle conseguenze derivanti da un elevato tasso alcolemico nel sangue mentre continuano a somministrare alcolici ai giovani, signor Ministro, è il parossismo dell'ipocrisia, è la cosa più inutile del mondo. Non avremmo biasimato un coinvolgimento attivo del Ministro della pubblica istruzione e delle politiche giovanili e avremmo apprezzato, per altri versi, anche un maggior impegno del Ministro dell'interno, soprattutto per un'efficace politica di controllo della rete stradale, partendo dalla necessità di mettere le Forze di polizia competenti nelle condizioni logistiche, ma soprattutto economiche, di operare con efficienza. Ci sono anche degli aspetti positivi in questo provvedimento. Noi crediamo che alla base di un provvedimento di questa natura ci debba essere tanto buon senso più che qualche fisima ideologica: il buon senso che ha portato il legislatore, in tempi recenti, ad imporre l'obbligo del casco, delle cinture, di un uso corretto dei cellulari in auto e così via. Questa politica dei piccoli ma determinanti passi ha portato ad un miglioramento delle statistiche incidentali ed è questo che mi fa pensare, in relazione al provvedimento che stiamo discutendo, ad un piccolo tassello di un mosaico che però è ben più ampio. Forse siamo ingenui ma prevenzione significa obbligare - signor Ministro, abbiamo discusso lungamente e nel dettaglio in Commissione circa questo problema - i ricchi enti gestori delle autostrade o proprietari delle strade a mantenere il manto stradale in perfette condizioni, a realizzare *guardrail* idonei, illuminazioni più potenti. Vi è un atteggiamento remissivo nei confronti dei potenti ed aggressivo nei confronti della gente comune, degli automobilisti. Non basta dire agli enti gestori, alle società concessionarie o agli enti proprietari delle strade di intervenire, ma bisogna dire che cosa succede se non lo fanno. Altrimenti credo - mi corregga se sbaglio - che l'articolo 24 sia assolutamente inutile.

perché non si vogliono obbligare quei soggetti a mantenere il manto stradale in perfette condizioni o a realizzare segnaletica orizzontale e verticale idonea o a illuminare sufficientemente le strade? Chi gira sulle strade europee vede altre cose: perché? Perché non aumentare i controlli incentivando le Forze di polizia e sollecitando una presenza più evidente sul territorio e sulle strade, rimpinguando gli organici dotandoli di attrezzature sofisticate? Sarebbe un controsenso non farlo e non approfittare di questa situazione perché chissà quando mai noi torneremo a discutere di sicurezza stradale. I controsensi di questa politica, signor Ministro, sono evidenti ed io ne cito alcuni che brillano nel testo e nella politica di questo Governo da alcuni mesi: Bersani che liberalizza le scuole guida elidendo di fatto un punto fermo nella formazione del giovane aspirante guidatore, mortificando le professionalità che pure c'erano e ci sono nelle scuole guida e poi il tentativo surrettizio, inserito nel testo, di recuperare quello sbaglio. Il ministro Turco che raddoppia la dose di *cannabis* per uso personale, fermata poi fortunatamente dalla giustizia amministrativa, e poi la richiesta di colpire, giustamente, chi guida sotto l'effetto di droghe. Sulla questione della velocità, signor Ministro, il problema non è riferito solo alla questione della droga e dell'alcol. L'articolo che modifica l'articolo 142 del codice dalla strada, che si occupa dell'osservanza dei limiti di velocità, è importante ma anche in questo caso il tratto distintivo del provvedimento è solo ed esclusivamente l'inasprimento delle sanzioni. Trovo ipocrita e anche un pò ridicolo consentire la costruzione di auto potentissime e poi stabilire sanzioni così pesanti sulla violazione dei limiti di velocità: visto che interveniamo sulla sicurezza delle auto occupiamoci allora anche di questo gravoso aspetto. Il codice della strada stabilisce limiti per tipo di strada, signor Ministro, per categoria di veicoli e quant'altro, ma consente agli enti proprietari, e io già in Commissione avevo richiamato la sua attenzione su questo delicato passaggio, la facoltà di fissare nuovi limiti, ovviamente inferiori e non superiori a quelli stabiliti dal codice della strada. L'ente proprietario deve occuparsi della posa in opera e anche della relativa segnaletica. Ci sono strade, però, ed anche tratti autostradali, dove il limite massimo è ridicolo e rischia di essere pericoloso: si rischia il tamponamento o di essere d'intralcio al traffico. Ma su quelle strade, su quei tratti autostradali vengono rilevate elettronicamente le velocità. Quanti sono gli automobilisti inutilmente colpiti e vessati, in questi casi? Non lo so, lo chiedo a lei, però sono numerosissimi, come si può vedere dal numero dei ricorsi. Anche la rimodulazione da tre a quattro fasce di misurazione dell'eccesso di velocità rappresenta un serio problema.

ma è comunque prevista la revoca della patente, che - come sappiamo - è uno strumento essenziale per milioni di italiani, che utilizzano la macchina per recarsi ad esempio al lavoro.

Questo è un vero ed autentico deterrente. E ciò non significa che io sostenga i frettolosi; sostengo invece il buonsenso, che mi fa notare come l'automobilista sia generalmente costretto nelle code, causate da un traffico intenso o dai lavori in corso, a velocità ridottissime. Abbiamo presentato qualche emendamento in Commissione e qualche altro lo abbiamo ripresentato in Aula, sperando che questi ultimi abbiano una diversa fortuna, che possano trovare un accoglimento da parte del relatore e del Governo, perché riteniamo che su un tema di questo genere sia veramente sciocco dividersi politicamente.

Presidente, i colleghi che ci hanno preceduto hanno già messo in evidenza l'anomalia di fronte alla quale ci troviamo, quella cioè di due provvedimenti

Questa è una tecnicalità a cui si ricorre per evitare il pericolo, come ha detto lA presidente Donati, che ci siano vuoti legislativi

al Ministro di avere seguito questo provvedimento con grande apertura, come ha sottolineato il senatore Filippi nella sua relazione. Ora, però,

Malgrado vari interventi legislativi, non siamo mai riusciti, se non nel caso della patente a punti, a ridurre in modo significativo questa vera e propria ecatombe, ecatombe, questa vera e propria emergenza nazionale. Cercherò di illustrare alcune riflessioni

provvedimenti sostanzialmente repressivi, senza allargare l'orizzonte ad una serie di cause che sono alla base di questa grandissima incidentalità. Non agiamo sui guidatori se non in misura molto modesta e, quindi, sull'educazione. Se in Aula sono stati presentati diversi ordini del giorno che vanno in questa direzione, in Commissione è emersa con grande forza la necessità di agire sotto il profilo culturale ed educativo nei confronti dei soggetti guidatori. Dobbiamo analizzare analizzare i vari elementi che concorrono all'incidentalità, la quale non si è ridotta malgrado i mezzi,

che qualche anno fa potevano essere mortali o comunque devastanti per i guidatori oggi sono totalmente neutri. Ciò vuol dire che i mezzi di locomozione e le stesse dotazioni per i guidatori sono molto più sicure rispetto al passato. Malgrado questo, però, non riusciamo a ridurre la mortalità e l'incidentalità in generale. generale. Dobbiamo pensare che una delle ragioni fondamentali è l'incremento del traffico circolante a parità di condizioni infrastrutturali.

Questo tema è di grandissima rilevanza proprio ai fini del risultato della sicurezza stradale. Inoltre, non abbiamo quasi mai, anzi direi che in questo provvedimento, ahimé, non ci sono, risorse adeguate per i controlli.

sicurezza stradale, che regoli la sicurezza della circolazione su strada, all'interno del quale possano riconoscersi e sentirsi rappresentati anche gli enti locali e le Regioni.

Dell'inadeguatezza delle infrastrutture abbiamo già parlato. Ricordo a me stesso, prima ancora che al Ministro e ai colleghi,

avere più di una vettura e, paradossalmente, nelle famiglie che non possono permettersele

con l'opposizione. È per questo che l'atteggiamento da parte nostra è stato e sarà anche in Aula estremamente costruttivo su questo provvedimento.

scippare due disegni di legge che alla fine sono finiti nel grande calderone: nel disegno di legge n. 1677, di cui parliamo, e una parte addirittura nella conversione del decreto-legge della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se fossero stati accolti nulla di grave nel senso che non è un problema di paternità. Sono stati così diluiti o sostanzialmente inapplicati che il problema posto dai due testi resta praticamente invariato. Il primo riguardava il problema della sicurezza stradale e, nello specifico, il problema giovanile che derivava dalla valutazione, di cui casualmente sono venuto a prendere atto, di ciò che l'ISTAT pubblica tutti gli anni: si registrano più di 200.000 incidenti mortali ogni anno che provocano più di 6500 decessi ed oltre 300.000 feriti. L'incidente stradale è considerato la prima causa di mortalità giovanile. È un dato assodato che non può lasciare il legislatore senza una reazione. Il testo presentato, che però non è stato recepito dall'assemblamento della Commissione, prevedeva una cosa diversa da quella passata: dei corsi specifici nel contesto della didattica scolastica. È importante conoscere l'italiano, come importante è conoscere la storia e come forse sarebbe altrettanto importante conoscere il latino che da tanto non si studia nelle nostre scuole. Però, è altrettanto importante imparare a vivere, imparare i comportamenti che poi avranno gli studenti da cittadini. Non vi è dubbio che da cittadino, tra le tante cose, si porrà, prima o dopo, alla guida di un veicolo, di un motociclo e così e così via. Il testo del Governo continua a parlare di educazione scolastica, come bastasse che i ragazzi conoscessero soltanto la cartellonistica stradale, che pure è importante;

i motocicli. Ciò che si chiedeva, e che non è stato recepito, è che ai ragazzi si insegni a scuola tutto quello che vuol dire prendere atto e la coscienza della guida di un mezzo a motore, con veri e propri corsi di guida. Non basta insegnare la cartellonistica. Al ragazzo bisogna dire che il motociclo è questo, la pista è una cosa e la strada è altro. guida con le ciabatte si rischia di lasciarci i piedi al momento che si ha un impatto e via dicendo. Ci sono organizzazioni del settore che girano, più o meno invitate *motu proprio*, cioè per iniziativa di qualche preside o di qualche

per chi commette altre violazioni. Per esempio, per chi guida con un tasso alcolemico superiore ad una certa soglia

Se, come corollario, dovessimo portare una serie di esempi passeremmo per i soliti razzisti. È però un dato statistico che tanti stranieri

però, secondo la norma del codice della strada, più severa del codice penale, oggi si rischia di più a uscire dal ristorante andando a casa senza provocare, non dico incidenti ma nessuna violazione o turbativa dell'ordine pubblico, che non guidando senza patente.

comminare per la guida con un tasso alcolemico assai alto è quella pecuniaria, che arriva fino a 12.000 euro.

A parte i costumi, a parte i modi di vita, probabilmente con due bicchieri di vino una persona non è incapace di intendere e volere, ma vogliamo paragonare o reprimere in modo più severo la persona che beve due bicchieri di vino rispetto a chi circola drogato fino ai capelli?

Pensavo di dare un piccolo contributo portando due norme che andavano a sanare due lacune che forse era meglio tamponare nel nostro ordinamento, usciamo con un testo che ha stravolto tutto e che sta inaugurando veramente l'era delle purghe, perché a questo punto un bicchiere di vino, una piccola violazione al codice della strada è considerata molto più grave di una violazione del codice penale: in Italia c'è qualcosa che non funziona.

che il tema della sicurezza stradale è uno di quei temi sui quali non dovrebbero esserci impostazioni ideologiche, ma sul quale dovrebbero svolgersi semplicemente delle considerazioni logiche

di cui si è parlato tante volte qui, anomalo ma necessario per permettere l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti, norme e disposizioni che erano indispensabili per aumentare la sicurezza nelle nostre strade, ed era importante farlo prima delle ferie, prima cioè del momento in cui si sarebbe avuta la massima punta della congestione del condizionamento veicolare sulla nostra rete.

esaminare, discutere e votare in Commissione e in Aula prima delle ferie, sono state fatte confluire nel decreto-legge del 3 agosto nella prospettiva, signor Ministro, lo sappiamo tutti, di un sua decadenza, e della volontà di trattare in quest'Aula complessivamente l'intero provvedimento; abbiamo saputo questa mattina che l'intenzione del Governo e della maggioranza non era questa,

possiamo oggi dire di essere compartecipi: le modifiche del codice penale, con l'inasprimento e la rimodulazione delle pene, anche amministrative,

pene più severe nei casi di guida senza patente, di eccesso di velocità, di uso del telefonino; divieto di trasportare su motocicli minori al di sotto di un certo limite di età e divieto, per tre anni, ai neopatentati di guidare motocicli o autovetture al di sopra di una data potenza; norme più stringenti sull'individuazione e l'informazione dei prodotti farmaceutici e poi altre norme a presidio dell'educazione stradale e contro l'inquinamento atmosferico e acustico, riportate nel disegno di legge. Un'ulteriore disposizione, introdotta a larga maggioranza in Commissione, conteneva la previsione di una pena accessoria, individuata nello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa in istituti ove sono ricoverate le vittime di incidenti stradali. Oggi constatiamo che il Governo e la maggioranza propongono un proprio emendamento soppressivo di tale norma, con la giustificazione che si tratta di una disposizione incostituzionale. Voglio dirlo subito (e lo ripeteremo durante la discussione): non siamo di questo parere; riteniamo che questa norma debba essere sostenuta e, comunque, nel caso così non possa essere, chiediamo al Ministro di farsene carico in ulteriori provvedimenti. Come ho detto, tuttavia, a conclusione dell'*iter* in Commissione, per le motivazioni suesposte, non siamo stati in grado di dare un voto positivo al provvedimento, ma abbiamo dovuto abbiamo dovuto esprimere una posizione di astensione. Esiste una fondata ragione su cui si basa tale scelta politica, che si ritrova nella convinzione che l'inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dal provvedimento e, naturalmente, l'effetto deterrente legato alla maggiore severità delle pene, non potrà produrre un innalzamento stabile delle condizioni di sicurezza sulle nostre strade, se non in presenza di una combinata azione di controllo e di repressione (azione di controllo e repressione che - è stato detto, ma lo devo ripetere ancora anch'io, perché credo che sia mio dovere - oggi è largamente insufficiente). Signor Ministro, nelle scorse settimane, ha dichiarato che nel primo semestre di quest'anno i controlli sulle strade sono stati raddoppiati

Bene, credo che queste iniziative vadano nella giusta direzione, ma la realtà è che tutto questo ci appare fortemente, incredibilmente inadeguato. Gli uomini, gli strumenti ed i mezzi attualmente a disposizione non bastano. Credo sia utile ricordare un dato che, personalmente, mi ha impressionato:

oggi, con oltre 35 milioni di veicoli, dei quali 5 milioni costituiti da mezzi pesanti, l'organico è rimasto lo stesso, la metà di cui il nostro Paese avrebbe bisogno.

dato ufficiale - è vetusto ed insicuro e molte auto hanno alle spalle diverse centinaia di migliaia di chilometri.

non può essere un fatto casuale che in Italia ci siano solo 170.000 controlli all'anno, mentre in Germania sono 5 milioni e in Francia 8 milioni.

teniamo presente che in Francia operano 1.500 *radar* installati sulla rete viaria e in Inghilterra ci sono 8.000 telecamere.

la riponga nel mettersi al passo con altri Paesi europei per quanto riguarda la dotazione di mezzi. Chiediamo al Governo, cioè, di mettere a disposizione degli organi di controllo mezzi e strumenti adeguati attraverso stanziamenti volti ad acquistare nuove tecnologie; penso ai *radar*, alle telecamere, all'ammodernamento dell'autoparco, alla revisione degli apparecchi e, se non sembrassi troppo minimalista, direi a stanziamenti che diano la garanzia anche della spesa corrente,

o di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze psicotrope o stupefacenti. Ripresenteremo le proposte emendative volte ad estendere l'obbligo in capo ai quattordicenni della patente di guida per condurre i ciclomotori e ad elevare l'età minima da 14 a 16 anni per la guida delle cosiddette

per coinvolgerli con i ministeri, le associazioni di categoria ed i privati nei programmi per la promozione e la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale con particolare riferimento ai rischi connessi alle sostanze alcoliche e stupefacenti. Un ultimo correttivo proposto si riferisce all'introduzione dell'obbligo normativo di accertamenti psico-diagnostici in sede di visita medica per il conseguimento della patente.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, l'incidentalità nei trasporti su strada rappresenta in Italia una vera e propria emergenza. Non sfugge pertanto l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti sottoposti al nostro esame aventi ad oggetto disposizioni volte ad incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Per avere un'idea del fenomeno, è sufficiente ricordare che l'incidentalità stradale rappresenta la nona causa di morte nel mondo e la prima nella popolazione italiana sotto i 40 anni. Le stime riportate dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti indicano che ogni giorno in Italia si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone ed il ferimento di altre I danni subiti dalle famiglie delle vittime sono enormi: il 90 per cento dei nuclei familiari di deceduti o vittime rimaste handicappate subisce una diminuzione della qualità della vita. Infatti, solo un terzo dei disabili torna a svolgere a tempo pieno il lavoro precedente. Il numero di anni di vita persi per incidenti stradali supera la somma degli anni persi a causa delle malattie cardiache e del cancro. Dal punto di vista economico essi sono responsabili di una perdita di circa il 2 per cento del PIL ed hanno un costo sociale che nel 2002 è stato quantificato in più di 34 miliardi di euro. È evidente, quindi, come questa delicata materia richiedesse un dibattito ampio ed esauriente che, seppur viziato dai tempi imposti dall'agenda parlamentare e dall'emergenza, è stato comunque possibile grazie alla sensibilità del ministro Bianchi verso il quale, anche a nome del gruppo della Rifondazione Comunista, intendo esprimere un sincero apprezzamento. L'Unione Europea e i singoli Stati membri, Italia compresa, hanno condiviso un obiettivo importante e impegnativo: il dimezzamento, entro il 2010, del numero delle vittime della strada. Ma secondo il rapporto di medio termine sul programma di sicurezza stradale europeo (Commissione europea, 22 febbraio 2006) l'obiettivo è ancora lontano e nonostante i progressi raggiunti, molto rimane da fare. L'approccio a queste tematiche deve a nostro avviso essere teso, da un lato, all'individuazione dei possibili interventi puntuali che sono propri della materia e che possono essere ricondotti sostanzialmente alla sfera preventiva, in particolare all'aumento dei controlli e alla riduzione dei limiti di velocità intraurbani, alla vigilanza rigorosa dei limiti di velocità; dall'altro, al decongestionamento del traffico veicolare nell'ottica di una mobilità sostenibile e pianificata che disincentivi così l'utilizzo del mezzo privato a vantaggio di quello pubblico. Sotto il primo profilo utili insegnamenti si possono trarre dalle esperienze condotte in altri Paesi europei; in particolare negli ultimi anni la Francia e l'Inghilterra hanno organizzato massicci controlli antialcol su strada nell'ordine di circa 5 milioni all'anno. Tali controlli hanno portato ad una notevole diminuzione delle morti, del 40 per cento in Francia e del 48 per cento in Inghilterra. In Italia vengono effettuati circa 3.900.000 controlli all'anno relativi a patenti libretti, a fronte di soli 200.000 o 500.000 controlli antialcol. Questo perché le pattuglie non hanno in dotazione etilometri.

Si tratta di un esempio emblematico che pure rende efficacemente l'idea delle misure che potrebbero essere, più di quelle penali, immediatamente introdotte e che potrebbero condurre da subito al conseguimento di significativi risultati, a fronte di una spesa che non risulterebbe neppure troppo gravosa. Occorre investire anche rispetto all'informazione: in Italia difatti si registra uno dei più bassi livelli di conoscenza del limite di alcolemia consentito alla guida, cento degli intervistati che afferma di non conoscerlo mentre il 4 per cento è convinto che sia superiore più del doppio del livello consentito. Occorre altresì evidenziare alcune contraddizioni in riferimento all'uso di alcol: da un lato, infatti, si interviene a livello di normazione primaria, dall'altro, sulla televisione e sulla stampa si registrano pubblicità che spesso veicolano modelli di vita e di comportamento consumistico che remano in senso contrario. Questa contraddizione riguarda anche la pubblicità di macchine sempre più veloci e sempre più potenti. Rispetto alla tematica dei controlli esprimiamo apprezzamento per quanto previsto dal disegno di legge, che destina un terzo delle maggiori entrate per il loro incremento. Per quanto riguarda il secondo profilo, la sicurezza stradale appare strettamente connessa con la problematica più generale della mobilità sostenibile. L'articolo 16 della Costituzione della Repubblica italiana recita che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, riconoscendo la mobilità e la possibilità di muoversi liberamente quale diritto fondamentale di cittadinanza. Il diritto alla mobilità deve essere, però, a sua volta, esplicitato con modalità capaci di garantire altri diritti, quali ad esempio il diritto all'aria pulita nelle città e nell'ambiente, alla sicurezza stradale dei cittadini, ad un ambiente urbano più vivibile, ricco di luoghi di incontro e con spazi pubblici di qualità elevata, cosicché tutto ciò non può essere messo in discussione dal diritto alla mobilità individuale, che pure deve essere garantito. Questo è quanto sta accadendo a causa dei grandi volumi di traffico nelle città e nelle autostrade: la libertà egoistica di ciascuno di spostarsi con mezzi privati sta erodendo lo spazio disponibile, la congestione veicolare aumenta, l'aria è sempre più inquinata, gli incidenti producono anche elevati costi economici e sociali e i diritti di ciascuno diminuiscono. Tali effetti producono una serie di costi non monetizzati dal sistema e costituiscono le cosiddette esternalità negative, ovvero costi prodotti da soggetti che dalle attività connesse con la mobilità traggono vantaggio ma che non pagano i danni che ricadono su terzi. Affrontare solo un aspetto delle problematiche derivanti dall'aumento del volume della mobilità delle persone e delle merci, intervenendo con accorgimenti puntuali sulla sicurezza delle strade e delle autostrade, sulla sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri, non è sufficiente se non si propone un diverso modello di mobilità basato sul trasporto pubblico delle persone e sul trasporto delle merci su rotaia e via mare in alternativa al trasporto su gomma, sul trasferimento di quote sul trasferimento di quote di traffico dalla gomma alla rotaia, sulla crescita delle strade del mare, sull'intermodalità, sul superamento della logica *tout court* delle grandi opere. È solo attraverso un approccio integrato alla mobilità che possiamo rendere davvero più sicure le nostre strade e le nostre autostrade. Infine, restano forti i temi che riguardano l'ingente aumento delle sanzioni amministrative e penali. Le nostre posizioni nel merito sono state già state espresse in Commissione, dove abbiamo manifestato la nostra perplessità rispetto alla loro forza deterrente. Il pericolo per noi, inoltre, è che si potessero introdurre degli elementi di soggettivismo che richiamano il diritto penale d'autore: «ti «ti punisco per come sei piuttosto che per ciò che hai fatto»; motivi di perplessità, questi, legati all'articolo 21 del disegno di legge che introduce delle aggravanti speciali ad efficacia speciale agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, cioè nei casi in cui il reato è commesso in condizioni di stato di ebbrezza o in caso di assunzione di sostanze psicotrope. Non si comprende, quindi, perché questa norma non sia stata estesa anche a coloro che superano i limiti di velocità previsti, avendo, essi, capacità logiche e coscienza attiva senz'altro superiori ai precedenti, consapevoli come siamo che il diritto penale, in quanto incide sulla libertà personale, che la Costituzione proclama inviolabile, deve limitare al massimo il suo intervento in una prospettiva di necessità di tutela anche del sistema penale. Non possiamo mai andare oltre una prospettiva di effettiva e concreta necessità della sanzione penale come estrema *ratio*. Occorre riconsiderare anche il fenomeno dell'etilismo in termini di problema sociale, andando nel fondo della questione, non più relegandola nella sfera delle scelte personali su come ci si intende svagare. Con le stesse considerazioni occorre riapprocciarsi al tema dell'utilizzo delle sostanze psicotrope: in entrambi i casi queste pratiche spesso derivano da disagi sociali a cui dovremmo prima o poi dare risposte. Riguardo all'uso di sostanze stupefacenti, c'è da fare un'altra considerazione: a differenza della guida in stato di ebbrezza, dove con l'etilometro si può dimostrare che effettivamente si è alla guida di un'automobile dopo aver assunto alcol, per quanto riguarda alcune sostanze - per esempio la *cannabis* - non ci sono strumenti o attrezzature per dimostrarlo. In alcuni casi i test sono sì capaci di individuare il consumo, ma non quando questo sia avvenuto, restando tracce fino a 90 giorni nel capello, 60 nelle urine, 30 nel sangue e 24 ore nella saliva. Occorre quindi per il futuro stabilire *standard* uniformi nell'effettuazione dei test antidroga, basati sull'evidenza scientifica, per individuare lo stato di alterazione psicofisica e non meramente il consumo passato, così come prevede il codice della strada. Sappiamo tutti quanto gli incidenti stradali agiscano sulla mortalità giovanile e qui esprimiamo un apprezzamento sia alla Commissione che al Ministro per aver accolto un emendamento che il Gruppo ha proposto per la soppressione dell'articolo 2, quello relativo alla guida accompagnata, perché sosteniamo che sia necessario prima lavorare sui modelli e sul comportamento alla guida, piuttosto che pensare sin da subito di creare un contesto di esercizio a tale pratica. Famose, purtroppo, sono le stragi del sabato sera e qui è fondamentale la ricostruzione - come vi dicevo - di modelli comportamentali e relazionali che abbiano la loro centralità nell'affermazione dell'essere sull'apparire. Bisogna sottrarre i nostri giovani alle logiche delle politiche consumistiche, non legare la loro realizzazione al raggiungimento di obiettivi sempre più legati alla materialità e alla sublimazione di *status symbol*. Onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Presidente, vorrei concludere con le considerazioni svolte da un ragazzo in un tema a scuola, il cui oggetto erano, appunto, le stragi del sabato sera, per indurre a riflettere che nella risoluzione dei problemi non si possono percorrere scorciatoie: «E contro la voglia di "sballare", "perdere il lume della ragione" e spesso "'autodistruggersi" del giovane cosa si può fare? Qui il discorso diventa più complesso, perché non ci sono divieti o controlli che tengano. Qui il problema sta alla radice, nell'insoddisfazione profonda dei giovani, che spesso sfocia in tentazioni suicide. Qui quello che manca, che forse la famiglia, la scuola, e in genere gli adulti non hanno saputo dare a questa nuova generazione, è il senso dell'esistenza, la certezza di essere voluti bene. Questo, secondo me, è il motivo profondo per cui un ventenne spinge l'acceleratore fino a rischiare la vita sua e dei suoi compagni di viaggio. Dietro l'apparente coraggio di chi vuole forse imitare i grandi piloti di formula uno c'è una grande insicurezza, un vuoto che tutti dobbiamo impegnarci a colmare».

Di questo bisogna dare atto per il lavoro svolto realmente ascoltando la voce del Parlamento, in particolare del Senato e della Commissione lavori pubblici, per cui va anche dato il giusto riconoscimento al relatore, al Presidente della Commissione e al Ministro che hanno dato la loro disponibilità su questo provvedimento. Vorrei sottolineare però alcuni punti riguardanti la sicurezza stradale in generale e, in particolare, in riferimento ad alcune norme che il provvedimento contiene. In questi casi, proprio per le norme approvate in linea di massima con il consenso generale, il rischio è l'eccesso di zelo, dell'emozione, anche più che comprensibile, causata da episodi recenti come le morti e i feriti causati da incidenti stradali che certamente bisogna fare ogni sforzo per ridurre. Gli eccessi di zelo sono sia quelli che possono essere contenuti nella legge, sia quelli che sono invece applicati in base alla segnaletica così come concretamente posta.

o per il traffico che ci può essere sulla strada stessa, allora è più che giusto, anzi è doveroso, il severo controllo per fare in modo che tali limiti siano rispettati

una tendenza di molti enti che hanno la responsabilità della segnaletica stradale - che, come sappiamo, sono in alcuni casi i Comuni, in altri le Province o i gestori delle autostrade - i

è? In generale gli automobilisti tendono a interpretare i limiti in questo modo, per cui quando c'è un limite posto come dovrebbe, cioè

senza curve, ad ampia visibilità e senza accessi «a raso», come si suol dire, rispettino effettivamente tale limite, perché infatti i limiti bisognerebbe rispettarli. Siccome però sappiamo che, nella realtà, questo vuol dire creare un intasamento, perché generalmente il limite viene interpretato come un eccesso di zelo, il risultato che abbiamo è, per certi versi, il mancato rispetto di limiti che invece andrebbero rispettati rigorosamente e per altri un rispetto di limiti che genera intralcio alla circolazione. Pertanto, innanzitutto, si genera un rallentamento, e non si può ignorare la libertà di spostamento dei cittadini, non dobbiamo ignorare che le strade servono a comunicare a non a rallentare i collegamenti tra un luogo e l'altro, e poi si crea una situazione di oggettivo pericolo perché di fronte ad un veicolo che, in situazione di piena visibilità, marcia a 40 chilometri all'ora in una strada su cui si potrebbe viaggiare senza problemi a 80 si crea si crea una coda dietro tale veicolo; dietro la coda arriverà qualcuno tentato di sorpassare, un sorpasso che potrebbe benissimo essere fatto in condizioni di sicurezza e che spesso è vietato, ma che trattandosi di colonna diventa pericoloso. Allora, io ho presentato due ordini del giorno: primo chiede al Governo di intraprendere un'azione, per quanto sia nelle sue possibilità, perché non è completamente nel potere del Governo la possibilità di intraprendere un'azione in questo senso, nei confronti dei gestori e di se stesso quando è direttamente il gestore, affinché i limiti di velocità ma anche i divieti di sorpasso e altri siano il più possibile sensati, siano il più possibile rigorosi e applicabili. Questo perché il rispetto della segnaletica, e della legge in generale, deve essere incoraggiato a verificarsi in modo puntuale e preciso.

lo credo. Penso che invece si dovrebbe fare un controllo il più possibile diffuso, anche severo, ma la severità può essere applicata solo a leggi e norme che siano realmente applicabili e non siano norme manifesto. A tale proposito, una semplice lettura del primo capitolo dei «Promessi sposi», dove si parla delle grida dell'allora governatorato spagnolo di Milano, dovrebbe illuminarci riguardo alle norme

velocità, ingresso in zona a traffico limitato nelle città, divieto di sosta e praticamente null'altro, a parte qualche multa per il passaggio con semaforo rosso riscontrato dai rilevatori automatici. Certamente, ci vuole una tutela, una disciplina, un rispetto di queste regole, ma le manovre spericolate, come il sorpasso a destra, il marciare contro mano e il sorpasso in zone dove si crea un reale pericolo,

Questo ricorso, però, è ammesso soltanto entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica stessa. Ciò ovviamente limita il diritto di coloro che hanno a che fare con tale segnaletica magari anche tre mesi o tre anni dopo che questa è stata apposta.

di rendere passibile di una multa il responsabile dell'apposizione della segnaletica dell'ente proprietario, che omette di rimuovere la segnaletica ad un pericolo o ad una situazione ormai passati. Il classico esempio è il cantiere o anche semplicemente il taglio dell'erba sul bordo della strada: si mette un bel limite di velocità di 20 chilometri

rettilineo ed un automobilista disciplinatamente rallenta, improvvisamente inchioda - come si suole dire - causando incidenti. Allora chi appone i cartelli deve ricordarsi di

dei trasporti*. Vorrei anzitutto dare atto dell'atteggiamento assolutamente costruttivo con cui si è svolta la discussione anche questa sera in Aula,

Farò quindi solo alcune brevi considerazioni in merito al percorso che ci ha portati fin qui stasera, anche per dire qualcosa a proposito del passaggio procedurale

che consideriamo di estrema gravità. Mi riferisco al numero di morti causato ogni anno dagli incidenti stradali, al numero di feriti, alle conseguenze di carattere economico, ad alcuni punti del prodotto interno lordo che sono il costo attribuibile agli incidenti stradali. In più sappiamo che questi incidenti sono in quantità superiore alla somma di quelli che avvengono sul lavoro, agli incidenti che avvengono per cause traumatiche (gli omicidi),

Sappiamo ancora - anche questo è stato richiamato poc'anzi - che l'incidente stradale rappresenta la prima causa di mortalità dei giovani.

di fronte alla quale ho promosso nei confronti del Governo un documento iniziale, tradottosi in un atto di indirizzo che il Governo stesso ha approvato alla fine di gennaio, in cui si poneva questa situazione nella sua crudezza - e non vogliamo dire drammaticità - e si proponeva una serie di interventi atti a contrastare detto fenomeno. Soggiungo come ulteriore elemento - anche questo è stato ampiamente richiamato - che la Comunità Europea si era data l'obiettivo di ridurre del 50 per cento l'incidentalità stradale entro il 2010

prendendo atto di tale condizione e per tutte le motivazioni che ho enunciato poc'anzi, l'atto di indirizzo presentato proponeva uno spettro molto ampio di interventi che potrei ricondurre a quattro linee di azione: sostanzialmente di formazione, d'informazione, di regole e di controlli. Queste sono le quattro linee sulle quali ritenevamo - e riteniamo tuttora - debba svilupparsi un'efficace azione

possa essere affidata solo al crearsi di una diversa cultura della sicurezza stradale, vale a dire del fatto di muoversi su una strada con un veicolo. Questa cultura ha dei tempi per formarsi, ma soprattutto deve partire dalle giovani e giovanissime generazioni. Sono perfettamente in linea con l'idea che, se l'educazione civica - peraltro, mi sembra anch'essa scomparsa dalle scuole contenesse al suo interno una parte relativa all'educazione stradale, avremmo fatto un passo in questa direzione. Nulla di simile è contenuto nel decreto-legge di cui stiamo discutendo, se non per cenni d'intenzione, perché nulla di simile era possibile

Ci è stato fatto rilevare che ciò comporterebbe una revisione complessiva dei programmi, un meccanismo un po' farraginoso; pertanto, abbiamo ripiegato e stiamo predisponendo, in raccordo

al giovane, o comunque alla persona che per la prima volta chiede di ottenere la patente, secondo me è inadeguata perché, nel migliore dei casi, quando venga fatta nel migliore dei modi,

Questo è un tema che riguarda la modifica dei programmi previsti per la formazione, svolti nella loro gran parte nelle autoscuole. Anche questo è un discorso aperto. Il secondo punto, come ho detto, è quello dell'informazione, che significa aprire più campagne di sensibilizzazione a questo tema. Abbiamo fatto una prima sortita qualche mese fa con una campagna radiofonica, altre ne stiamo predisponendo. Credo che su questa strada dovremmo non fermarci più: alimentare cioè continuamente l'informazione nei confronti dell'utenza, preferibilmente e possibilmente selezionandola, (per esempio, per i giovani stiamo curando particolarmente il segmento della scuola), perché appunto vi sia attenzione a questo fenomeno e alle conseguenze che comporta. Il terzo Programma nazionale per la sicurezza stradale, quello finanziato con la legge finanziaria 2007, sta puntando esattamente in questa direzione

informare il guidatore nel momento in cui sta sulla strada, perché un guidatore informato delle condizioni ambientali nelle quali si trova, delle modifiche che questo ambiente può subire nel tempo, informato sulle condizioni della strada, sugli incidenti presenti, sui lavori,

con la segnaletica, di cui ha parlato poc'anzi il senatore Malan (e tornerò sull'aspetto che egli ha sottolineato), ma ha molto a che vedere con la possibilità di utilizzare la telematica per una informazione interattiva e continua nel tempo. Dobbiamo cioè, sia con segnalatori luminosi sulle strade a messaggio variabile e con il rinvio anche in auto di messaggi, fare in modo che appunto guidatore sia costantemente informato di quello che lo circonda. Non vi è spazio anche per questo tipo di attività nel provvedimento, c'è spazio ampio negli negli atti che stiamo via via perfezionando in attuazione del Programma nazionale della sicurezza stradale. Dico questo perché vorrei sottolineare l'importanza di portare avanti

provvedimento assolutamente essenziale per migliorare lo stato della prevenzione e della sicurezza stradale e che, tuttavia, nell'arco di poco tempo, di tre anni di applicazione, ha esaurito quasi completamente la sua efficacia. La riduzione in un triennio è stata notevolissima: circa il 20 per cento degli incidenti in meno; ma di questa riduzione, il 90 per cento si è concentrato quasi tutto nel primo anno e mezzo. Il che significa, in buona sostanza, che questo provvedimento ha avuto una sua fisiologica caduta di efficacia (che era anche normale aspettarsi: dopo aver dispiegato tutti i suoi effetti assieme, è venuto un po' meno) e, in secondo luogo, che si sono sviluppati una serie di meccanismi reattivi da parte degli utenti della strada, che, ad esempio, sanno meglio come evitare l'autovelox, fino ad arrivare a comportamenti meno dignitosi, come quello di attribuire i punti persi ad un parente prossimo, ricordato in più occasioni. Una recente statistica ci racconta che una che una percentuale impressionante di punti sono attributi a persone che hanno più di 80 anni di età, il che significa che ci stiamo attrezzando alla bisogna. Poi c'è un altro meccanismo di cui ci siamo resi conto da poco e che dobbiamo contrastare: l'eccessiva facilità con cui questi punti vengono restituiti.

al quale abbiamo molto creduto e lavorato sotto forma di disegno di legge, a un certo punto si è posta la necessità e l'opportunità, alla fine di luglio, di trasformarlo in un decreto-legge, affinché nel periodo periodo di maggior traffico e maggior numero di incidenti, come avviene ogni anno, si potesse disporre di alcune norme di base efficaci: sei articoli che puntavano agli aspetti più delicati. Non posso dire adesso che questi abbiano prodotto chissà quali effetti nel mese di agosto, anche perché non disponiamo di dati statistici, però sicuramente abbiamo proseguito nella creazione di un'atmosfera di attenzione e controllo verso questo fenomeno. Ora la nostra intenzione, come ho esplicitamente detto all'inizio dei lavori in Commissione trasporti, è quella di lavorare sul disegno di legge. A noi interessa portare a termine il disegno di legge, anche perché questo contiene ben altro che il decreto‑legge.

decreto per una ragione qualsiasi, non dipendente nemmeno dalla nostra volontà, dalla volontà dell'Aula o dallo sviluppo della discussione, avrebbe infatti creato un danno grave, soprattutto, come è stato ricordato prima anche dal senatore Cicolani, per tutti gli aspetti di carattere penale contenuti nel decreto si sarebbe prodotto un vuoto che avrebbe creato un grave *vulnus* nell'amministrazione della materia. Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di accondiscendere alla richiesta, che abbiamo trasferito in Commissione, di approvare il decreto così com'è, in modo secco, quindi senza intervenire in nessun modo Abbiamo pertanto scelto in Commissione trasporti di non emendarlo e di

La seduta è tolta